Chiedo che tutto ciò venga acquisito come testimonianza dell'estrema nobiltà del collega Forte per aver fatto parte di quest'Assemblea, nel momento in cui da tanta parte di essa si riteneva che la giustizia avesse giustamente esercitato i suoi poteri criminali nei confronti di parlamentari italiani, ad onore del fatto che l'UDC aveva deciso di candidare il collega Forte nell'altra legislatura e per il fatto che questa assoluzione, da noi lungamente attesa, giunge molto, troppo tardi. Già altre volte, troppo tardi sono stati prosciolti, perché il fatto non sussiste e non solo per non averlo commesso, personaggi ed esponenti della politica locale, regionale e nazionale dell'allora mio partito, la Democrazia Cristiana, e non soltanto di quel partito, a testimonianza del fatto che su queste vicende il Ministro della giustizia dovrebbe riferire, altro che le proposte che intende fare nella legislatura:

per quel tipo di processo che anche in quest'Aula troppe volte è stato richiamato contro ipotetici corrotti e corruttori. Mai come in questo caso, mai come nel caso del senatore Forte, il solo fatto che il sindaco Forte fosse stato arrestato mentre era ricoverato in clinica per un intervento chirurgico, tredici anni dopo, lo assolve, perché il fatto non sussiste. del senatore Forte, dico ciò in questo momento e chiedo che il Senato tutto pronunci la condanna per questa vergognosa abitudine della magistratura italiana di tenere sotto processo anni una persona e chiudere, al termine dell'indagine dibattimentale, dicendo che il fatto non sussiste. C'è da chiedersi quali fossero i magistrati che all'epoca avevano chiesto il processo

ha prospettato un'ipotesi di riforma, stabilendo dei tempi (non so se anche per il processo penale, ma ne dubito) per il processo civile. Gli posso fare tanti auguri, ma credo che situazioni del genere non possano essere risolte con dei pannicelli caldi. Occorre una nuova cultura del diritto e della giustizia. Se non la si acquisisce i casi Forte, come tanti altri che ad esso somigliano, diventeranno sempre diventeranno sempre più numerosi e più gravi. Non auguro a nessuno di capitare nel tritacarne giudiziario, ma purtroppo questo tritacarne è così efficiente anche a causa dei tempi dei processi penali. prossimi saranno giorni di riflessione, vi saranno le inaugurazioni dell'anno giudiziario: credo spetti alla politica cominciare a dare risposte serie, non guardando in faccia a nessuno. una nuova finestra"). Do comunicazione delle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo che, riunitasi questa mattina, ha approvato all'unanimità il nuovo calendario dei lavori fino al 1° febbraio 2007. Come già previsto, la seduta pomeridiana di oggi sarà dedicata allo svolgimento di interpellanze e interrogazioni. Nella seduta antimeridiana di domani, mercoledì 24 gennaio, verrà discussa la mozione n. 48 con procedimento abbreviato, di iniziativa dei senatori Pisanu ed altri, sui rapporti tra Italia e Libia. La votazione di tale mozione avverrà in apertura della seduta pomeridiana, con inizio alle ore 16. A seguire, sempre domani pomeriggio, il ministro Mastella svolgerà la relazione sull'amministrazione della giustizia, prevista dalla nuova legge sull'ordinamento giudiziario, alla quale seguirà un dibattito per complessive tre ore e trenta minuti, ripartite tra i Gruppi. Sono escluse dal contingentamento le dichiarazioni di voto sulle eventuali proposte di risoluzione che saranno votate a conclusione della seduta. A tal fine, la seduta stessa potrà protrarsi oltre l'orario consueto. Nella seduta antimeridiana di giovedì 25 gennaio saranno poste all'ordine del giorno interpellanze e interrogazioni. La prossima settimana, nel pomeriggio di martedì 30 gennaio sarà discussa la modifica dell'articolo 5 del Regolamento, per la cui votazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Seguirà l'esame di due documenti in materia di insindacabilità. Nella seduta antimeridiana di mercoledì 31 gennaio sarà posto all'ordine del giorno, ove concluso dalla Commissione, il decreto-legge recante abrogazione di una norma su illeciti contabili, per il quale si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi. Nella seduta pomeridiana dello stesso giorno saranno discusse le dimissioni presentate dal senatore a vita Francesco Cossiga. Proseguirà poi, eventualmente, l'esame del decreto-legge citato. Nella seduta antimeridiana di giovedì 1° febbraio saranno esaminate le mozioni e gli altri strumenti presentati sulla questione dell'ampliamento della base USA di Vicenza. Nel pomeriggio avrà luogo il sindacato ispettivo. Infine, il calendario potrà essere integrato con la deliberazione dell'Assemblea per la costituzione in giudizio in un conflitto di attribuzioni. **Programma dei lavori

non vi è alcun dubbio che, come è stato più volte affermato, il rilancio della pubblica amministrazione non possa realizzarsi se non attraverso una strutturata e complessiva politica di valorizzazione delle risorse umane. Se, infatti, si intende veramente rendere la pubblica amministrazione motore dello sviluppo economico e del rilancio del «sistema Italia», non si può prescindere dalla effettiva valorizzazione delle tante professionalità, competenze e risorse, quotidianamente impegnate nel fornire servizi efficienti ed efficaci ai cittadini e all'intero sistema produttivo. A tal fine il Governo sta già lavorando per dare adeguate risposte attraverso un radicale rinnovamento della formazione professionale, delle retribuzioni salariali, della riprogettazione informatica delle procedure, nonché tramite lo snellimento di farraginosi *iter* che determinano un duplice danno, sia di funzionalità e di efficienza verso gli utenti che di immagine nei confronti dell'amministrazione stessa. In tal senso, infatti, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Consiglio dei ministri del 1° dicembre, previo parere favorevole della Conferenza unificata, ha definitivamente approvato il disegno di legge recante norme sulla modernizzazione e la semplificazione della pubblica amministrazione che presto inizierà la sua strada di approvazione in Parlamento. Lo sforzo compiuto per garantire il rinnovo dei contratti del pubblico impiego per il biennio 2006-2007, contenuto nella stessa legge finanziaria 2007, nonché la stabilizzazione dei lavoratori precari, completa il quadro di un impegno serio e stringente del Governo per far fronte alle esigenze della pubblica amministrazione. Tanto rilevato, in risposta, senatore Sacconi, alla sua interrogazione, non risulta che «i dirigenti che si occupano di personale e relazioni sindacali vengono nominati solo dopo aver sentito le organizzazioni sindacali» o che il «direttore dell'Ufficio relazioni sindacali del Dipartimento della funzione pubblica (...) dovrà essere designato dalle organizzazioni sindacali». In particolare, senatore Sacconi, per quanto attiene quest'ultimo rilievo, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ha individuato un dirigente del Dipartimento della funzione pubblica, referendario dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, in possesso di una qualificata professionalità e di una specifica esperienza nel settore, maturata presso gli uffici dello stesso Dipartimento; lo stesso, infatti, ha svolto per diversi anni la propria attività, prima come funzionario e poi come dirigente, presso l'Ufficio relazioni sindacali e presso l'Ufficio del personale delle pubbliche amministrazioni del suddetto Dipartimento; il cosiddetto ufficio UPPA, che il senatore Sacconi conosce molto bene. Per quanto riguarda la questione relativa alla presidenza dell'ARAN, occorre, in via preliminare, precisare quanto segue. Come è noto, il comitato direttivo della stessa agenzia è costituito da cinque componenti, compreso il presidente, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Di questi, due componenti sono designati da soggetti estranei al Governo (uno dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e l'altro dall'ANCI e dall'UPI congiuntamente). Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia, designa, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città, gli altri tre componenti, tra i quali il Presidente. Al momento dell'insediamento del nuovo Governo, il comitato direttivo dell'ARAN, nominato con un decreto presidenziale del 20 marzo 2006, risultava composto soltanto dai tre componenti designati dall'Esecutivo, in quanto la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e le associazioni degli enti locali non avevano indicato alcun nominativo. Peraltro, il presidente del comitato, che all'atto della designazione rivestiva l'incarico di Capo di Gabinetto dell'allora Ministro per la funzione pubblica, era stato nominato nonostante, in data 1° marzo 2006, in sede di parere della Conferenza unificata, le Regioni avessero espresso a maggioranza parere negativo - e altrettanto avesse fatto in precedenza l'UPI motivando lo stesso, non sulla base di un giudizio negativo nei confronti del soggetto designato, ma in considerazione delle specifiche competenze richieste dall'incarico. A ciò si aggiunga che la nomina del presidente e dei componenti del comitato è stata effettuata ben oltre la data di scioglimento delle Camere, ovvero nel periodo sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 2002, n. 145. Pertanto, risulta di tutta evidenza che tale assetto incompleto del comitato non ha potuto assicurare lo svolgimento delle attività dell'organismo stesso, in particolare nella delicata fase di avvio delle trattative relative ai rinnovi contrattuali per il quadriennio 2006-2009. Al fine, quindi, di assicurare la piena operatività dell'Agenzia attraverso la ricostituzione ed integrazione del comitato, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto del 15 novembre 2006, ha provveduto, ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 luglio 2002, n. 145, alla revoca del presidente uscente e di un componente del comitato direttivo, rispettivamente il consigliere Raffaele Perna e il signor Edoardo Calzoletti. Inoltre, il Comitato direttivo non era, comunque, nella possibilità di funzionare per effetto delle dimissioni presentate dall'altro componente, dottor Guida, tenendo conto che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento generale di organizzazione dell'ARAN, per le riunioni del medesimo comitato è necessaria la presenza di almeno tre componenti. Successivamente, nelle more della ricostituzione del Comitato ed al fine di garantire la funzionalità dell'ARAN, si è proceduto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 novembre 2006, a nominare l'avvocato Massimo Massella Ducci Teri commissario straordinario dell'Agenzia; ciò in considerazione della particolare professionalità e della specifica competenza acquisite dallo stesso nel corso del suo precedente incarico di componente del medesimo Comitato. Infine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2006, il comitato è stato integralmente ricostituito con le modalità e sulla base delle designazioni acquisite ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei requisiti professionali ivi indicati. In tale ambito, l'avvocato Massella è stato nominato presidente del comitato direttivo, previo parere favorevole della Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città, espresso all'unanimità. Per quanto riguarda, inoltre, il caso del direttore dell'Ufficio per gli affari generali ed il personale, iscritto ad una organizzazione sindacale fin dal 1974, si ricorda che l'attuale incarico gli è stato conferito dal precedente Governo esclusivamente sulla base, ne siamo tutti convinti, dei suoi requisiti professionali. In merito all'ultimo punto della sua interrogazione, senatore Sacconi, si fa presente che il Governo, nel mettere mano alla riorganizzazione della pubblica amministrazione e degli apparati organizzativi, intende perseguire, tra gli obiettivi principali, proprio quello di garantire l'eliminazione di ogni possibile conflitto di interesse.

che il nuovo Governo avrebbe avviato una politica di cogestione con le organizzazioni sindacali delle amministrazioni pubbliche, determinando in esse ulteriore inefficienza attraverso l'esaltazione dei vizi già presenti, quali innanzitutto la irresponsabilità di tutti gli attori, dalla direzione politica alla dirigenza, al diffuso mondo del pubblico impiego. Invero, le informazioni che mi sono state fornite sono incomplete o non corrispondenti alla verità dei fatti: due membri dell'ARAN sono diretta espressione di due organizzazioni confederali sindacali e gli altri sono - potremmo dire - collaterali ad esse. Il Capo del personale del suo Ministero è contemporaneamente il responsabile dell'area dirigenziale di una grande confederazione sindacale in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, cui appartiene la sua stessa amministrazione. Non è in discussione la qualità delle persone, molte delle quali conosco anche personalmente e stimo, ma la linea che voi praticate nello scegliere queste persone o nel consentire ad esse lo svolgimento contemporaneo

divinò quanto poi sarebbe accaduto. Voi conferite alle organizzazioni sindacali e alla contrattazione poteri di organizzazione che sono sempre rimasti nell'autonoma disponibilità del datore di lavoro nel settore privato e della funzione politica come della dirigenza nel settore pubblico, perché vi impegnate a condividere con le organizzazioni sindacali la scelta dei settori e delle attività *non* *core*, cioè ancillari a quelle istituzionali, da esternalizzare. Vi impegnate a concordare la mobilità, che può essere solo contrattata o volontaria. Concordate gli accessi, al punto che stabilizzate, comunque e dovunque siano, anche in sedi già eccedentarie, a prescindere quindi dall'esigenza delle amministrazioni, i circa 300.000 cosiddetti precari. Concordate con le organizzazioni sindacali l'accesso alla dirigenza per progressione verticale, probabilmente consentendo implicitamente anche il consenso o il veto sindacale alla scelta degli stessi dirigenti che per progressione verticale si determineranno. Vi impegnate a concordare con il sindacato perfino i sistemi di valutazione e di sanzione della dirigenza e dei suoi uffici. Insomma, siamo davvero ai *soviet*. Siamo davvero a organismi cogestionali che delegittimano definitivamente la dirigenza pubblica. Contemporaneamente, proprio dalle vostre fila sorge una proposta di legge (che qualche incauto mio collega di opposizione ha firmato alla Camera, mi auguro che nessuno al Senato vorrà seguirlo) in ordine all'istituzione di una nuova Autorità per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, dimenticando che l'autorità c'è (e probabilmente merita di essere riformata) ed è la Corte dei conti, ma soprattutto che la valutazione dei meriti e dei demeriti nelle amministrazioni pubbliche tocca alla dirigenza e questa non deve essere delegittimata, per un verso consegnandola nelle mani di un'impropria cogestione con il sindacato e per altro verso sottoponendola ad una nuova Autorità indipendente di valutazione solo perché lo consiglia il "Corriere della Sera" attraverso il professor Ichino. Penso che abbiate preso la strada peggiore per rimettere ordine nelle amministrazioni pubbliche; se fannulloni ci sono, e certamente ci sono, oltre a persone straordinariamente meritevoli, voi incoraggiate i primi e demotivate i meritevoli.

come evidenziato dal senatore Manzione, si propone di realizzare in via sperimentale un servizio pilota per la raccolta e la gestione centralizzata delle chiamate di emergenza. Ciò al fine di consentire ai cittadini, in qualunque Stato europeo essi si trovino, di attivare i competenti servizi di soccorso nazionali chiamando un numero unico, il 112. Considerato che le infrastrutture di telecomunicazione costituiscono un'irrinunciabile opportunità tecnologica per gestire in modo efficace ed immediato immediato le situazioni emergenziali, le istituzioni europee hanno voluto promuovere l'introduzione del numero unico 112 nelle reti telefoniche pubbliche degli Stati membri, pur nella dichiarata consapevolezza delle difficoltà che le amministrazioni nazionali avrebbero incontrato nel coordinare ed implementare le specifiche misure organizzative esistenti in ciascun Paese. Se, da un lato, infatti, al cittadino europeo è riconosciuta la possibilità di utilizzare una sola numerazione per segnalare qualsiasi tipo di emergenza, dall'altro, all'amministrazione è imposto l'onere di raccogliere le segnalazioni, di analizzarle e di indirizzarle ai diversi enti che dovranno gestirle a livello operativo (Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco, In attuazione delle prescrizioni comunitarie, nel corso della precedente legislatura, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2003, è stata avviata la fase propedeutica all'attivazione sul territorio nazionale di questo innovativo servizio. In particolare, è stato costituito, presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle diverse amministrazioni interessate. A tale gruppo di lavoro è stato assegnato il compito di realizzare uno studio per l'analisi delle problematiche connesse all'avvio della sperimentazione e di definire, quindi, un piano di attuazione e di coordinamento delle conseguenti iniziative. A seguito dell'approvazione dello studio di fattibilità del progetto, avvenuta nel marzo 2005, è stata, poi, costituita una struttura di missione denominata «Unità tecnico-operativa per l'istituzione del numero unico europeo di emergenza» con il compito di definire, organizzare e coordinare le attività necessarie all'attuazione del progetto, fornendo, altresì ai soggetti attuatori gli opportuni indirizzi amministrativi, organizzativi e tecnici. Inoltre, in attuazione dell'articolo 127, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il numero unico europeo di emergenza è stato individuato, con decreto del Ministro delle comunicazioni, quale servizio abilitato a ricevere le chiamate di emergenza provenienti dalle numerazioni 112, 113, 115 e 118. In seguito, e fino al termine della scorsa legislatura, la sperimentazione del numero unico si è, tuttavia, bloccata a causa di problematiche organizzative e tecniche che l'attuale Governo si sta impegnando a superare per dare rinnovato impulso all'attuazione del progetto. Le maggiori difficoltà operative derivano, in particolare, dalla circostanza che l'avvio del progetto richiede il coinvolgimento di una pluralità di istituzioni pubbliche, centrali e locali, ai fini della necessaria integrazione delle tecnologie informatiche di *hardware* e *software*, telefoniche e radiofoniche, attualmente utilizzate dai singoli centri operativi di Carabinieri, Polizia e Vigili del fuoco. In tal senso, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ha avviato una proficua collaborazione con il Ministero dell'interno e con il Ministero delle comunicazioni che ha già prodotto un importante risultato. Il progetto è stato profondamente modificato rispetto all'impostazione data nella precedente legislatura. Si è ritenuto, infatti, di non procedere alla fase sperimentale ed all'attuazione di un *call center* di primo livello, ma di prevedere un unico numero di emergenza gestito dalle centrali operative già esistenti. Mi riferisco alle sale operative di Polizia di Stato, Carabinieri e Vigili del fuoco, che costituiscono il primo terminale per le segnalazioni di emergenza. Ciò consentirà di ridurre significativamente i costi di avviamento e di formazione del personale, in quanto si prevede di utilizzare operatori già da tempo qualificati nella gestione delle emergenze. Tale scelta operativa consente, inoltre, di ridurre sia i tempi di realizzazione del progetto sia quelli di intervento per la gestione coordinata delle emergenze, a vantaggio della collettività. Dunque, l'avvalersi di personale e di strutture già esistenti e qualificate rende possibile evitare un'ulteriore fase di sperimentazione e avviare la fase operativa del progetto entro la fine del 2007. Infine, per quanto concerne il finanziamento già ottenuto, pari a 9.700.000 euro, destinato a consentire l'avvio della sperimentazione nelle province di Salerno, Palermo e Catanzaro, lo stesso risulta confermato e verrà utilizzato per provvedere all'estensione a regime del progetto in questione. Il Governo, quindi, consapevole della rilevante importanza della realizzazione del numero unico di emergenza, intende recuperare i ritardi registratisi finora nell'attuazione del progetto e dare risposta, in tal modo, alle contestazioni della Commissione europea.

a quella che potremmo definire una mancata attuazione dell'impegno comunitario, rispetto al quale l'Italia aveva assunto degli obblighi precisi. Condivido tutta la sua ricostruzione, collega, tranne l'ultima parte. Noi dovremmo avere il coraggio di chiamare sempre le cose con il loro nome: non possiamo raccontare alla gente che esiste una differenza sostanziale, di DNA, tra chi agisce sempre nell'interesse generale e chi invece, a volte, riesce a piegare l'interesse generale per fare in modo che quantomeno coincida con interessi particolari. Quel che voglio dire che ci trovavamo di fronte alla realizzazione di un progetto ambizioso ed importante. Era importante perché, come ha detto lei molto correttamente, realizzava degli obiettivi che dovrebbero appartenere a quel sistema di ammodernamento del Paese

dovevamo riconoscere, come è giusto fare, che il centro-destra aveva avviato in maniera corretta un percorso che - lo ribadisco, è bene dirlo quando ciò coincide con la verità - era riuscito ad avvicinarsi alla soluzione del problema. Ha ragione lei quando dice che bisogna vincere delle resistenze e che bisogna integrare delle amministrazioni molto diverse, ma il senso di questo progetto era proprio vincere questa grande battaglia che portava ad una centrale unica per l'emergenza

che le specificità e le diversità, che nelle rispettive amministrazioni molto spesso determinano problematiche non facilmente risolvibili, fossero affrontate all'interno di questo organismo e fossero risolte, se è vero com'è vero che si era arrivati già alla fase della sperimentazione; se è vero com'è vero che poi si era attraverso questo gruppo, a un *memorandum* d'intesa con il commissario Reding per l'estensione del progetto anche al tema della sicurezza stradale. E guardi, sottosegretario Magnolfi, che che la ricostruzione che propongo, e che voglio resti agli atti per fare in modo che non tutti pensino che si è capaci di mistificare la realtà a proprio piacere,

alle contestazioni che venivano fatte a livello europeo alla procedura d'infrazione n. 2006/2114, specificava come in effetti tutto fosse stato ripristinato, tranne quel gruppo interministeriale che è stato smantellato perché purtroppo non sempre noi recuperiamo la serietà e la capacità di leggere in filigrana e di comprendere che ci sono organismi tecnici che devono continuare un lavoro che hanno messo in campo.

proprio perché occorreva ragionare in questa direzione, era stata prevista una sperimentazione che, nell'affermazione in risposta all'infrazione fatta dal nostro Governo, veniva indicata essere

«metteremo invece a regime il progetto nel 2007» non venivano ritenute soddisfacenti dall'Unione Europea, se è vero com'è vero che veniva notificato, il successivo 18 ottobre, l'elaborato formale con il quale veniva emesso un parere motivato proprio relativamente alla contestazione d'infrazione che io indicavo. l'Europa ci contesta; noi sosteniamo che comunque realizzeremo nei tempi la sperimentazione che sarà nel 2006 limitata ad una sola Provincia e a regime nel 2007; adesso, invece, sottosegretario Magnolfi, lei viene qui - siamo nel 2007 - a dirci una cosa diversa da quello che lo stesso Governo, un mese e mezzo fa, ha riferito all'Unione Europea. Non penso di potermi dichiarare soddisfatto. Evidentemente c'è stato qualcuno che ha voluto affermare una logica muscolare per la quale tutto quello che fanno gli altri va distrutto. Non si fa così nel Governo, bisogna essere capaci - lo dicevo prima - di guardare in filigrana e di comprendere quali sono i meccanismi automatici che stanno realizzando interessi generali, e che vanno quindi tutelati, e quali sono invece le realtà rispetto alle quali il Governo legittimamente debba intervenire. Si è persa una grande occasione per dimostrare che c'è una diversità di DNA. Evidentemente, quando si governa, quando si comanda, molto spesso le differenze non esistono e c'è solo la necessità di occupare il potere. Questo è un caso specifico di occupazione ingiusta di potere e di ritardo di un sistema di ammodernamento del Paese, che chiaramente graverà sulla Provincia di Salerno e sull'Italia tutta. *(Applausi del

Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, questa nostra interpellanza prende le mosse da una delle pagine più drammatiche della storia militare del nostro Paese, nonché da una delle vicende più significative della nostra storia contemporanea. Prende le mosse dal settembre 1943, da Cefalonia. Una vicenda che ha inizio nel luglio del 1940, quando Mussolini decise quella campagna d'aggressione della Grecia che, nel volgere di poche settimane, si trasformò in una *débâcle*, l'ennesima rovinosa esperienza del colonialismo italiano. La storia ci ricorda che l'alleato nazista intervenne in soccorso della fallimentare impresa italiana; la Wehrmacht riuscì ad occupare Atene e le isole ioniche, tra cui Corfù e Cefalonia, affidando il controllo militare di queste ultime al presidio della Divisione italiana Acqui del generale Gandin. L'8 settembre 1943 venne ufficializzato l'armistizio con gli anglo-americani. Quella stessa sera giunse a Cefalonia, dalla sede di Atene del comando misto italo-tedesco, un comunicato firmato dal generale Vecchiarelli di sostanziale conferma del proclama di Badoglio. Ma la sera seguente il generale Vecchiarelli, costretto dai nazisti, smentì l'ordine precedente e disconobbe il patto siglato dal generale Badoglio. A Gandin, come agli altri comandanti di divisione, venne impartito l'ordine di cedere le armi ai tedeschi e di trasferire alla Wehrmacht il controllo del territorio. Nei giorni seguenti accadde quell'episodio che, il 10 marzo 2001, il presidente della Repubblica Ciampi - rompendo la «congiura del silenzio su Cefalonia», come ebbe a definirla vent'anni prima Pertini definì essere una delle pagine più gloriose della Resistenza italiana. La Divisione Acqui, rifiutando le ingiunzioni di subordinazione di Vecchiarelli e l'*ultimatum* tedesco dell'11 settembre, decise, in seguito ad un *referendum* interno, di non consegnare le armi e di dare il via alla resistenza antinazista. Resistenza che prese forma in un dolorosissimo scontro militare al termine del quale caddero in battaglia 1.200 soldati italiani. La preponderanza delle forze di terra e di cielo tedesche indusse il generale Gandin a decidere la resa. Il 22 settembre, giorno in cui la resa fu comunicata al nemico, l'esercito nazista fece scattare una caccia all'uomo nei confronti dei militari italiani. 155 ufficiali e 4.500 soldati italiani vennero catturati, fatti prigionieri e massacrati, in violazione dei codici internazionali di guerra e di qualsiasi convenzione militare. Cosa hanno a che fare questi fatti, acquisiti alla memoria storica, con la cronaca di questi mesi e, dunque, con la nostra interpellanza? Nel luglio 2006 a Monaco di Baviera si è concluso il primo grado del processo ai danni di Otmar Mühlhauser, uno dei protagonisti reo confessi dell'eccidio, al tempo comandante del plotone di esecuzione che passò per le armi numerosi ufficiali italiani della Divisione Acqui. August Stern, procuratore generale del tribunale di Monaco, ha disposto il proscioglimento dell'ex sottotenente tedesco e, quindi, l'archiviazione del processo. Nella sua ordinanza, il procuratore sostiene che i militari della Divisione Acqui erano da considerarsi «traditori paragonabili a disertori», vigliacchi voltagabbana schieratisi dalla parte del nemico («nemici combattenti») e quindi indegni del riconoscimento e del trattamento di prigionieri di guerra. Per Stern l'omicidio colposo - che pure egli è costretto a riconoscere - è privo delle «circostanze aggravanti» e quindi il reato cade in prescrizione. Dal momento che il codice penale tedesco definisce «omicidio colposo aggravato ogni omicidio commesso nei confronti di una persona [...] per avidità o ulteriori vili motivi», l'assenza delle aggravanti indica che Stern non ha reputato «vili» i motivi che hanno spinto Mühlhauser a ordinare la fucilazione degli italiani. Le motivazioni dei militari tedeschi non erano vili - ha sostenuto nelle scorse settimane Stern, cercando goffamente di difendere la propria sconcertante tesi giudiziaria - perché essi non le ritenevano tali. Capite bene, signor Presidente, signor Sottosegretario, che ciò significa, sul piano storico e giuridico, attenuare, se non addirittura giustificare e legittimare, le responsabilità di coloro i quali compirono quel tremendo eccidio. Significa accettare in pieno il punto di vista, e quindi le ragioni, dei criminali nazisti. L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia lo ha dichiarato esplicitamente, stigmatizzando l'ordinanza di Stern «in nome dei princìpi di libertà e giustizia ai quali si è ispirata la lotta per Liberazione nel nostro Paese, nel più vasto quadro della lotta dei popoli liberi per la democrazia e la giustizia». Visto che la corte penale di Monaco, nella persona dello stesso procuratore Stern, è chiamata nelle prossime settimane a giudicare sul ricorso che la figlia di una delle vittime di Cefalonia ha presentato contro la decisione di prescrivere il reato al signor Mühlhauser, in questo contesto chiediamo al Governo di considerare tutta la gravità della situazione. Noi riteniamo che questa non sia e non possa essere più considerata una vicenda giudiziaria normale e, dunque, di ordine privato. Riteniamo che siano in causa, oltre alla memoria, anche la dignità e l'onore di combattenti italiani che sono stati vittime di condotte inammissibili e che, per ciò che effettivamente è avvenuto, meritano un riconoscimento formale ed istituzionale. Non si tratta, a nostro modo di vedere, di giudicare un comportamento e nemmeno vorrei chiarirlo, perché ci è stato contestato - di interferire con la giustizia tedesca, con la magistratura di un altro Paese che ha la sua autonomia e la sua indipendenza. D'altra parte l'insigne parere consegnatoci dal professor Giuliano Vassalli, ex presidente della Corte costituzionale, ci pare essere, in tal senso, una garanzia. Ciò che vorremmo, e chiediamo al Governo se non lo ritenga opportuno, è che vengano fatti passi ufficiali perché si determini una presa di posizione istituzionale, da parte del nostro Paese, affinché la Germania, in tutte le sue articolazioni istituzionali, riconosca la verità storica e dia alla verità storica, in questo caso quella dei massacri perpetrati dai militari nazisti, la dovuta diffusione, la dovuta visibilità e ciò suoni come esplicito riconoscimento e scuse nei confronti dei nostri militari. Chiediamo, in definitiva, che il Governo italiano ottenga dal Governo tedesco il netto riconoscimento dell'indegnità dell'ordinanza e, per questa via, della verità storica. Una verità storica che è - come è stato detto - incompatibile con le argomentazioni contenute nel dispositivo di archiviazione. Una verità che nessun revisionismo potrà modificare. Viviamo una fase segnata da continui tentativi di riscrivere la storia, cercando ignobilmente di portare sul banco degli imputati non già gli aguzzini nazisti e fascisti ma coloro i quali hanno combattuto per la libertà e per la democrazia. Le 6.000 vittime di Cefalonia e le centinaia di migliaia di vittime del nazifascismo ci ricordano ogni giorno che esistono torti e ragioni immodificabili.

il Governo concorda pienamente con l'onorevole interpellante sulla inaccettabilità delle motivazioni dell'ordinanza con cui la procura di Monaco ha disposto l'archiviazione del procedimento penale contro l'ex ufficiale dell'esercito tedesco, Otmar Mühlhauser, uno dei responsabili della fucilazione dei militari italiani a Cefalonia nel settembre del 1943. Appena informati dell'ordinanza, tramite il nostro ambasciatore a Berlino, abbiamo espresso immediatamente al ministro federale della giustizia, Brigitte ed al ministro della giustizia della Baviera, Merk, la nostra indignazione e deplorazione per le tesi del procuratore di Monaco, ribadendo l'importanza di ristabilire la verità storica e giuridica e richiamando anche, al riguardo, la condanna erogata dal tribunale di Norimberga contro il generale Hubert Lanz, comandante delle truppe tedesche a Cefalonia. Nella circostanza, abbiamo altresì tenuto a sottolineare alle autorità tedesche che quella di Cefalonia è una pagina gloriosa della storia italiana, rammentando il numero dei militari italiani caduti sotto il fuoco tedesco per tenere fede al loro giuramento di fedeltà alle istituzioni nazionali italiane. Tali argomentazioni sono state ribadite in successivi incontri con questo ambasciatore di Germania e con autorità tedesche a Berlino. Le risposte non si sono fatte attendere. In una lettera al nostro ambasciatore a Berlino, il ministro della giustizia della Baviera, Merk, ha dato atto che «il massacro compiuto contro i soldati italiani a Cefalonia ha infranto, in maniera terrificante e disonorevole» - sono le parole del Ministro - «le regole del diritto internazionale di guerra». Lo stesso Ministro ha aggiunto che «è altrettanto fuori discussione che non vi era alcuna giustificazione per quelle azioni. Pertanto, con l'archiviazione del procedimento, la procura di Monaco non ha assolutamente voluto mettere in dubbio quanto affermato al momento della condanna del generale Hubert Lanz nell'ambito dei processi di Norimberga sulle fucilazioni di Cefalonia». A questa inequivocabile presa di posizione sull'aspetto politico e storico della vicenda, il ministro Merk fa seguire un'articolata ricostruzione tecnico‑giuridica del dispositivo della sentenza. Riassumerò qui gli aspetti principali evocati dal ministro Merk. Primo: nell'ordinanza della procura di Monaco non vi è nessuna intenzione assolutoria. È fuori di dubbio - come lo stesso pubblico ministero Stern ha tenuto a precisare per iscritto - che «al comportamento dell'indagato non può essere riservata comprensione alcuna»; secondo: il termine «traditori» nel dispositivo dell'ordinanza della procura di Monaco era virgolettato; esso non si riferiva infatti all'operato delle forze armate italiane, ma alla percezione che, all'epoca, il sottotenente accusato aveva degli avvenimenti. Nelle parole del ministro Merk «l'indagato avrebbe dovuto comprendere che i militari italiani rimanevano fedeli alla propria Patria, ma nella sua ottica soggettiva egli percepiva quei soldati, che prima erano stati compagni d'armi, come nemici che lottavano contro di lui»; terzo: questa percezione - sottolinea il ministro Merk - era sicuramente sbagliata e inaccettabile tanto dal punto di vista giuridico, quanto da quello morale. Tuttavia, il fatto che l'accusato abbia agito, a suo tempo, per obbedire ad ordini ricevuti e sulla base di una comprensione distorta della realtà fa sì che nei suoi confronti non scattino oggi le aggravanti previste dal codice penale tedesco per l'omicidio doloso aggravato per «vili ragioni». Non è quindi, sul piano strettamente tecnico, erroneo ammettere che i reati contestati all'imputato possano cadere in prescrizione. Ai fini di una valutazione della lettera del Ministro della giustizia bavarese, riteniamo che le argomentazioni giuridiche a sostegno della decisione di archiviazione da parte della procura di Monaco vadano tenute distinte dalle considerazioni di carattere storico e morale sulla vicenda di Cefalonia e sul comportamento dei militari italiani. Se sul piano giuridico risulta insoddisfacente la giustificazione ricercata nelle interpretazioni giurisprudenziali invocate nel caso Mühlhauser, dal punto di vista del giudizio sostanziale, la lettera rappresenta una chiara presa di distanza tanto del Ministro tanto del Ministro quanto dello stesso pubblico Ministero rispetto a quella che appariva come un'offesa della verità storica, della dignità delle vittime della tragedia di Cefalonia e delle Forze Armate italiane. Sotto questo profilo, i passi svolti con le autorità tedesche sono riusciti nell'intento di ottenere, da parte delle medesime, una precisazione inequivocabile sul comportamento dei nostri militari: i propositi del ministro Merk e del procuratore generale non avrebbero

Signor Presidente, colleghi, ringrazio il Sottosegretario per la risposta che, tuttavia, ritengo solo parzialmente soddisfacente. Vorrei che si tenesse tutti conto di un fatto oggettivo che dovrebbe indurci a leggere questa vicenda sotto una prospettiva diversa rispetto a quella - mi si consenta di definirla parziale - assunta nella risposta. Il fatto oggettivo indiscutibile è che il procedimento a carico del criminale di guerra nazista Mühlhauser è ancora in corso; si è concluso soltanto il primo grado di giudizio. Questo significa - lo ribadisco - che la presa di posizione da parte dello Stato italiano può e deve essere forte, netta ed impegnativa. Sappiamo bene che uno Stato non può costituirsi parte civile in un processo. Non chiediamo ciò che sul piano della procedura giuridica non è possibile. Chiediamo invece che singole persone, esponenti autorevoli delle istituzioni del nostro Paese, rappresentino la comunità nazionale italiana in quel procedimento. Se è vero che quell'ordinanza di archiviazione ha infangato la dignità delle vittime e ha tentato di stravolgere la verità storica, come anche lei ha riconosciuto, allora è del tutto evidente che è urgente e necessaria una presa di posizione delle istituzioni italiane attraverso cui opporsi, con estrema chiarezza, a quello scempio e a quel tentativo di riscrivere la nostra storia. Non vogliamo certo aprire una crisi diplomatica con la Germania. Siamo convinti, al contrario, che le istituzioni di quel Paese, nate dal ripudio della tragedia nazista, non possano che essere al nostro fianco. Dobbiamo intervenire, dunque, e rendere pubblica una questione che, sino ad oggi, abbiamo l'impressione si sia risolta in un fatto privato tra la signora De Negri, parte civile italiana, e il procuratore Stern, che ha espresso il giudizio ed ordinato l'archiviazione. Prova del fatto che questa vicenda è rimasta, sino ad ora, privata sono anche le informazioni da lei presentateci, che solo oggi diventano di dominio pubblico.

La signora De Negri, che sinora a proprie spese ha svolto questo importante ruolo, non può e non deve essere lasciata sola. conclusione, vorrei aggiungere un'ulteriore considerazione su cui credo valga la pena riflettere. È un dato di riflessione storica. La giustizia tedesca non ha mai, fino ad oggi, condannato alcun militare della Wehrmacht o delle SS resosi responsabile di assassinio, massacro e violenza nei confronti di militari italiani. Non vi è mai stata una condanna. Anzi: ogni qualvolta un'autorità giudiziaria tedesca abbia, per incidenza nel contesto di un procedimento penale, emesso una sentenza in tal senso, la Corte suprema ha sistematicamente provveduto a prescrivere o ad assolvere. Ci pare, dunque, che l'episodio oggetto dell'interpellanza, si inserisca in un contesto più ampio e quantomeno problematico. L'intervento equilibrato, ma inequivocabile e fermo - delle nostre istituzioni dimostrerebbe, proprio in ragione di questo contesto, che il nostro Paese vuole dare un contributo reale, in termini di conoscenza e di verità storica, in modo da rifuggire da qualsiasi forma di revisionismo storico. Ce lo chiedono i militari di Cefalonia e coloro i quali negli anni bui del nazismo e del fascismo, pagando anche con la vita, hanno scelto di lottare per la libertà.

Signor Presidente, onorevoli senatori, la vicenda cui fa riferimento l'interrogazione si ricollega all'indagine che ha portato, il 15 novembre scorso, all'esecuzione di misure di custodia cautelare nei confronti del sindaco e di un assessore del Comune di Montesilvano, indagati per i reati di corruzione aggravata in concorso ed associazione per delinquere, nonché di alcuni imprenditori e dipendenti dell'ente locale. L'inchiesta riguarda il conferimento di lavori pubblici alla ditta Green Service, il cui amministratore era già stato precedentemente arrestato. Gli sviluppi di altre due *tranches* investigative riguardanti la medesima vicenda hanno successivamente portato all'emissione di un secondo provvedimento di custodia cautelare nei confronti dello stesso sindaco, notificato in carcere l'11 dicembre, ed all'arresto di un altro assessore, indagato per i reati di concussione e calunnia. A seguito dell'operazione richiamata nell'interrogazione, peraltro, già il 20 novembre scorso la maggioranza assoluta dei consiglieri comunali aveva rassegnato le dimissioni contestuali dalla carica determinando così una delle fattispecie di scioglimento del Consiglio comunale previste dal testo unico sugli enti locali. Conseguentemente, il prefetto di Pescara ha disposto la sospensione del Consiglio comunale e la nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente, avviando la procedura di scioglimento degli organi elettivi che si è poi perfezionata con decreto del Presidente della Repubblica del 12 gennaio 2007. Al momento dell'operazione del 15 novembre, la notizia degli arresti degli amministratori di Montesilvano ha avuto vasta eco in ambito locale e regionale, attirando l'attenzione degli organi d'informazione, che in quell'occasione hanno quindi rivolto numerose domande al questore di Pescara. Rispondendo alle sollecitazioni dei giornalisti, il questore ha dichiarato che l'operazione non era ancora conclusa, che ci sarebbero stati sviluppi e che durante le indagini si erano registrate pressioni diffamatorie nei confronti del dirigente della Squadra mobile allo scopo di farlo estromettere dall'incarico. Tale circostanza risulta confermata anche dalle notizie acquisite dal Ministero della giustizia presso la procura della Repubblica di Pescara. In particolare, si è appreso che, dopo che era stata conosciuta l'esistenza di indagini in corso, il dirigente della Squadra mobile è stato fatto oggetto di calunnie e diffamazioni che tendevano a ledere la sua onorabilità ed a far supporre un suo accanimento nei confronti degli indagati per motivi personali. Il procuratore della Repubblica, portato a conoscenza di tali circostanze, ha riconfermato piena fiducia al dirigente della Squadra mobile e, insieme al sostituto assegnatario del fascicolo, ha fatto in modo che le indagini procedessero senza intralcio. Della vicenda e della sua evoluzione lo stesso questore ha tenuto informata la Direzione centrale anticrimine del Dipartimento di pubblica sicurezza. Successivamente, i responsabili delle pressioni lamentate sono stati individuati e denunciati all'autorità giudiziaria, davanti alla quale pende ora procedimento penale per calunnia a carico di tre persone nei cui confronti è stata chiesta ed ottenuta la custodia cautelare in carcere anche per questo reato. Nel rispetto per le attività in corso da parte della magistratura, ritengo opportuno che il Governo si astenga dal formulare considerazioni sulla vicenda finché essa non sarà stata definita in sede giudiziaria. Quel che si può dire sin d'ora, comunque, è che i fatti così come descritti dimostrano che è stato fatto tutto il possibile sia per garantire la funzionalità dell'ente locale, sia per tutelare la serenità, l'indipendenza ed il lavoro dei funzionari impegnati nella delicata inchiesta.

Io, sul punto della vicenda, ho formulato questa interrogazione perché ritenevo importante che venisse in qualche modo dato atto ai funzionari dello Stato che sono andati avanti nel perseguire i presunti responsabili - perché naturalmente siamo ancora a livello di istruttoria, anche se caratterizzata da esecuzione di provvedimenti di custodia cautelare - della loro correttezza e della loro, direi, fedeltà allo spirito di servizio che dovrebbe sempre contraddistinguerli e mi sembra che il Governo sia consapevole di questo. Ci auguriamo che questi riconoscimenti siano sempre più frequenti, anche maggiormente testimoniati di fronte all'opinione pubblica. Voglio approfittare di questa circostanza perché queste vicende, secondo me, al di là del caso particolare, interessano, naturalmente, una massa enorme di amministrazioni locali, sono anche determinate da un insufficiente ordinamento degli Enti locali. So che il Governo ha elaborato e presenterà un disegno di legge su questo tema. Io mi chiedo, lo chiedo a me stesso, chiedo a lei, signor Sottosegretario, lo chiedo al Governo ed ai colleghi, se non occorra sin da subito ripensare ad un sistema di controlli sull'attività degli Enti locali che, tra l'altro, è presente per le attività delle amministrazioni centrali, pensiamo alla Corte dei conti, al Consiglio di Stato e così via, ma è carente per gli Enti locali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione. Io credo che occorra ripensare a questa situazione di compatibilità costituzionale, di controlli e di nuovo quadro costituzionale perché, senza i controlli, vicende quali quella che si è manifestata a Montesilvano, che purtroppo potrebbero manifestarsi in tanti Comuni, in tante Province, sono destinate

dell'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, prima di rispondere all'interrogazione del senatore Brutti, desidero innanzi tutto esprimere la mia personale solidarietà e quella del Governo al sostituto procuratore presso la Direzione distrettuale antimafia di Napoli, magistrato particolarmente impegnato nei confronti di indagini contro organizzazioni di tipo mafioso nel casertano, così come a tutte le persone soggette a minacce per il loro quotidiano impegno al servizio dello Stato. Posso assicurare, per quanto riguarda le misure per la sicurezza personale adottate nei confronti del sostituto procuratore, che l'esposizione a rischio del predetto è stata sempre oggetto di approfondita valutazione da parte della Prefettura di Napoli. Detto ufficio territoriale del Governo, nel corso degli anni, ha costantemente rimodulato il dispositivo di protezione, incrementando le misure di tutela indicate nello specifico decreto ministeriale del 28 maggio 2003, in relazione all'entità del rischio. La prefettura di Caserta ha disposto l'attuazione di adeguate misure di vigilanza in occasione della presenza in Provincia del predetto magistrato. Ovviamente, come comprenderà bene il senatore Brutti, non posso scendere in dettagli ma vi sono misure di vigilanza anche nei confronti dei familiari. Per quanto riguarda invece le minacce nei confronti della giornalista del quotidiano «Il Mattino», queste risalgono a diverso tempo fa e non sembrano essere collegate alla conclusione del cosiddetto processo Spartacus. In relazione a questo ultimo evento sono state, viceversa, attuate misure di protezione nei confronti del presidente del collegio giudicante e di un componente la II sezione della corte d'assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Ricordo, altresì, che lo scrittore da lei citato fruisce di uno specifico servizio di tutela, a cura dell'Arma dei carabinieri, disposto in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in data 16 ottobre 2006. Misure di protezione individuali sono state attivate e, successivamente intensificate, anche nei confronti dell'ex parlamentare, già segretario della Commissione parlamentare antimafia, in seguito a dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, secondo cui il predetto esponente politico sarebbe un possibile obiettivo della criminalità organizzata, nonché per il rinvenimento di scritte minacciose nei suoi confronti. Comunico, infine, per completezza di informazione, che sono stati attivati dispositivi di protezione, commisurati al livello di rischio, nei confronti di altri diciotto magistrati che svolgono il proprio incarico istituzionale in Campania. Circa le iniziative per debellare le organizzazioni malavitose, è noto che nella provincia di Caserta agisce il *clan* camorristico denominato dei Casalesi, che estende la propria influenza ben oltre i confini dei paesi d'origine, in modo da formare un vero e proprio «cartello criminale» ramificato nel territorio. Il sodalizio criminale è strutturato, infatti, secondo un rigido e complesso sistema oligarchico di controllo, da cui dipendono vari referenti zonali, scelti dal vertice malavitoso per la gestione delle attività illecite nelle diverse aree. Il nucleo storico dell'organizzazione è costituito dalle famiglie Schiavone-Bidognetti-Iovine-Zagaria, i cui vincoli parentali danno al gruppo una notevole capacità di rigenerazione. L'attività di contrasto dispiegata sul territorio casertano da parte delle forze dell'ordine è costantemente mantenuta a livelli sempre molto elevati, anche in considerazione della crescente domanda di sicurezza della collettività. Dal gennaio 2005 ad oggi, sono state condotte a termine numerose operazioni di polizia giudiziaria, che hanno consentito la cattura di alcuni esponenti di spicco dell'organizzazione criminale e di assicurare alla giustizia un centinaio di affiliati del clan. Nel 2006 le forze di polizia hanno tratto in arresto 20 pericolosi latitanti e, il 23 dicembre 2006, sono state arrestate 15 persone, accusate a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso. All'inizio del corrente anno 17 persone, accusate a vario titolo di associazione mafiosa, sono state arrestate ed altre 16 indagate in stato di libertà. In particolare, nello scorso anno sono stati arrestati tre elementi di spicco del clan dei Casalesi, uno del clan Mazzacane ed un elemento di vertice del sodalizio Mazzoni inserito nell'elenco dei primi 500 ricercati in campo nazionale. Tale intenso e costante impegno investigativo, che non ha precedenti nei confronti del crimine organizzato casertano, è confluito in complessi procedimenti penali, celebrati dinanzi la corte di assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere - tra cui anche quello ricordato dall'interrogante - a conclusione dei quali sono state inflitte numerose, pesanti condanne. Nonostante ciò, il sodalizio criminale dei Casalesi conserva ancora la propria capacità operativa, in quanto risultano tuttora latitanti alcuni personaggi di primo piano dell'organizzazione, due dei quali inseriti nell'elenco dei 30 ricercati più pericolosi d'Italia. Al riguardo, il questore di Caserta ha assicurato che la ricerca dei latitanti è una priorità assoluta dell'azione investigativa della questura e delle altre forze di polizia, proprio in considerazione della loro pericolosità derivante dal forte potere di aggregazione che i medesimi sono in grado di esercitare nei confronti degli altri appartenenti all'organizzazione criminale. Per quanto riguarda l'attività della Direzione investigativa antimafia di Napoli, comunico che sono in corso diverse iniziative di contrasto al crimine organizzato presente nella Provincia, sia nell'ambito del coordinamento delle indagini di polizia giudiziaria, sia in quello, di provata efficacia, di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, che colpiscono direttamente - come è noto - gli interessi economici della criminalità. In questo campo nel corso del 2006 sono stati sequestrati ad appartenenti al *clan* dei Casalesi beni per un complessivo ammontare di oltre 16 milioni di euro. Analogo impegno viene profuso dalle forze di polizia nel contrasto della criminalità diffusa che, nella Provincia, si manifesta principalmente nella città di Aversa e nei centri limitrofi con reati di tipo predatorio. in quanto tale fenomeno delinquenziale, oltre a produrre anch'esso allarme sociale, costituisce un importante serbatoio per il reclutamento di delinquenti comuni da parte delle cosche successivamente impiegati in reati ben più gravi rispetto ai danni di persone e di beni. Il solo commissariato di Aversa, nel corso di servizi di controllo del territorio, nel corso del 2006, ha tratto in arresto in flagranza di reato 80 persone. Ricordo, inoltre, che già dal 2004, le riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica (C.P.O.S.P.) sono state estese, oltre che ai Sindaci dei Comuni interessati, anche ai rappresentanti delle associazioni di categoria dei commercianti e degli imprenditori. Ciò al fine di approfondire la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica, soprattutto in relazione ad episodi intimidatori commessi ai danni di appartenenti a dette categorie. Allo scopo di diffondere la cultura della «sicurezza partecipata», anche per meglio contrastare il fenomeno delle estorsioni, è stata chiesta la collaborazione dei cittadini e delle stesse vittime, invitando i Sindaci dei maggiori Comuni della Provincia, tra cui Aversa, a promuovere incontri mirati, nel corso dei quali rappresentanti della prefettura e delle Forze di polizia hanno illustrato i benefici derivanti dall'applicazione della normativa antiracket ed antiusura e le modalità più opportune per l'attuazione di misure di protezione passiva. Sempre in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, è stato approntato un piano coordinato di controlli nei confronti di esercizi pubblici, siti in Casal di Principe e in Parete, che sono gestiti o abitualmente frequentati da soggetti collegati alla criminalità organizzata. Ciò per l'eventuale adozione, in caso di riscontro di irregolarità, di provvedimenti sanzionatori, finalizzati a prevenire più gravi illeciti. Le forze di polizia, coordinate in sede di Comitato, vengono continuamente impiegate in capillari servizi di controllo del territorio sia con il personale dei locali presidi territoriali, sia con i rinforzi provenienti da altri reparti. A tal fine, nel corso del 2006, il Comando Regione Carabinieri ha potenziato il dispositivo nell'agro-aversano assegnando complessivamente 25 nuove unità a supporto dei reparti territoriali ed, in particolare, dall'8 maggio del 2006 sono state assegnate 10 unità al Gruppo Carabinieri di Aversa e, dal successivo 16 ottobre, ulteriori 15 unità sono state destinate ai Comandi Compagnia di Mondragone e di Casal di Principe. Per la parte di competenza, la Prefettura segue attentamente le attività delle amministrazioni comunali sotto il profilo del pericolo di infiltrazioni mafiose. A tale proposito, ricordo che nella Provincia di Caserta sono stati sciolti i consigli comunali di San Tammaro e Casaluce, mentre è ancora in corso l'attività delle commissioni d'accesso per gli accertamenti ai sensi della normativa antimafia presso i Comuni di Casapesenna, Castel Volturno, San Cipriano d'Aversa, Marcianise e Lusciano. [BRUTTI

mi dichiaro soddisfatto delle sue risposte all'interrogazione presentata. Vorrei sottolineare alcuni aspetti delle affermazioni che abbiamo appena ascoltato da parte del vice ministro Minniti, perché mi sembrano politicamente significativi per definire qual è il piano dell'azione di contrasto alle organizzazioni camorristiche in un territorio come quello della Provincia di Caserta. presenta, infatti, alcune peculiarità che la distinguono rispetto ad altre aree di insediamento camorristico. Qui abbiamo un'organizzazione centralizzata in un territorio ristretto; essa rassomiglia non tanto alle articolate cosche della camorra della Provincia di Napoli, all'interno delle quali abbiamo assistito in questi anni,

Ha una struttura difficilmente penetrabile, ha un vertice, dei capi, ha capacità di penetrazione nelle istituzioni. L'elenco, che il vice ministro Minniti ci proponeva, dei Comuni per i quali è stato disposto l'accesso e sono in corso accertamenti ai fini della decisione circa un possibile scioglimento delle amministrazioni fa riferimento a Comuni già segnati da una lunga storia di penetrazione camorristica, di compromissioni con i gruppi criminali, di dominio della criminalità organizzata. L'azione dello Stato c'è.

i processi, i dibattimenti, i giudizi si fanno presso i tribunali. E il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha scarse forze, ha un'organizzazione limitata, ha risorse non sufficienti

Le minacce di azioni ritorsive e le intimidazioni cominciano nel dicembre 2005, dopo la sentenza di condanna del processo denominato Spartacus, ove furono condannati tutti i capi del *clan* dei casalesi. Da lì partono le minacce in più direzioni, soprattutto ai giudici ed è da apprezzare il riferimento analitico che qui il rappresentante del Governo ha fatto ai magistrati che, dopo quelle intimidazioni, sono stati messi in una condizione di protezione e di tutela. Minacce gravi sono state poi rivolte ad un nostro compagno, un parlamentare dei Democratici di Sinistra, impegnato in prima linea nella lotta contro la camorra. Voglio dire al rappresentante del Governo che l'ultima drammatica peculiarità della camorra casertana è che la sua organizzazione centralistica fa capo a due *clan* e a due capi. I due capi della camorra casertana sono Francesco Schiavone e Francesco Bidognetti, entrambi, signor Presidente, in carcere; entrambi sottoposti ad un regime carcerario severo; entrambi sottoposti all'applicazione dell'articolo 41-*bis*. E, nonostante questo, essi, dall'interno del carcere, continuano a dirigere l'organizzazione camorristica nella Provincia di Caserta. Ciò pone due problemi: luogo, l'azione anticamorra deve essere più forte sul terreno dell'aggressione ai beni ed ai capitali che sono nella disponibilità delle organizzazioni camorristiche, perché il prestigio di quei capi, che sono in carcere, deriva dal fatto di poter continuare a gestire affari ed a manovrare capitali; luogo, l'applicazione concreta dell'articolo 41-*bis*, le condizioni concrete di vita carceraria dei capimafia e dei capicamorra. Consegno all'attenzione del rappresentante del Governo questo tema di riflessione che credo debba essere fatto proprio anche dalla Commissione antimafia e debba rappresentare un punto di riferimento dell'azione di contrasto alla quale tutte le istituzioni sono chiamate per sconfiggere le organizzazioni mafiose.

Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero innanzitutto cogliere l'occasione per rinnovare in questa sede, ancora una volta, l'apprezzamento e la gratitudine a tutti gli investigatori ed operatori di polizia che hanno contribuito in vario modo alla cattura di Bernardo Provenzano, conseguendo così un importantissimo e lungamente atteso successo nella lotta alla criminalità organizzata. Penso così di interpretare anche la volontà del Parlamento. Come riferisce la Questura di Palermo, l'operazione che ha portato all'arresto di Provenzano si è svolta la mattina dell'11 aprile scorso intorno alle ore 11, quando personale della Polizia di Stato ha catturato il *boss* latitante in una masseria in località Montagna dei Cavalli, nelle campagne di Corleone. Oltre a Provenzano, nell'operazione è stato arrestato anche, per favoreggiamento personale, il proprietario della masseria; immediatamente dopo, sono stati avviati sul posto i rilievi tecnico-scientifici e le altre necessarie attività d'indagine. La notizia della cattura, come evidenziato nell'interrogazione, risulta essere stata diffusa circa mezz'ora dopo, cioè a distanza di un lasso di tempo minimo e comunque strettamente necessario ad informare le autorità competenti. Lo stesso giorno, il Ministro dell'interno *pro tempore* ha poi tenuto una conferenza-stampa al Viminale assieme al Procuratore nazionale antimafia, al Capo della Polizia ed ai Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Dagli elementi in nostro possesso, quindi, non sussistono motivi per ritenere che fra la cattura di Provenzano e la formale comunicazione della notizia all'opinione pubblica sia intercorso un lasso di tempo significativo.

associamo al sentimento di stima e di apprezzamento nei confronti delle forze dell'ordine. È un sentimento di apprezzamento e di stima, signor Vice ministro, che manteniamo nel tempo, non ondivago, a seconda delle manifestazioni cui partecipiamo. Sicuramente non la sua parte politica, ma altre forze non manifestano gli stessi sentimenti o comportamenti di apprezzamento

Un dubbio che ci viene, ma che possiamo cogliere magari anche nel *web,* é però da quanto tempo fossimo pronti ad arrestarlo. È un dubbio legittimo che ci poniamo. Sono tempi molto ristretti, tempi forse del politicamente corretto, ma il dubbio che l'arresto sia stato in qualche modo ritardato per non intervenire nel confronto elettorale lei oggi non lo ha in alcun modo dissipato. Se allora è pensabile che quell'arresto sia stato in qualche modo fatto disinnescare qualche giorno dopo, rimane un dubbio:

la macchina del Ministero dell'interno in qualche linea di comando non abbia avuto l'ordine di aspettare che si calmasse la *kermesse* elettorale. Questo sarebbe molto grave: sarebbe stato un

liste. Anche in questo caso, l'interpretazione è sempre stata politicamente corretta, ma a sinistra. Lasciamo questi interrogativi, non facciamo sensazionalismo come Deaglio,

che forse qualche altro disegno potesse essere ipotizzabile, che forse la vittoria già annunciata del centro-sinistra poteva essere condivisa da qualcuno all'interno della catena di comando.